gentili senatori, evidenzio preliminarmente che l'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 71 del 2024 ha previsto, esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025, la possibilità di utilizzare, entro il 31 dicembre 2024, le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, al fine del raggiungimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I vincitori dei concorsi scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi disponibili prima delle nomine a tempo determinato, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 99, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi. La norma prevede, altresì, che i docenti eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024-2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima Regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto e che, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali, i posti vacanti resi disponibili sono coperti mediante contratti a tempo determinato sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie d'istituto. La norma richiamata, dunque, prevede inequivocabilmente la conferma per gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi, di cui ai decreti direttoriali 2575 e 2576 del 2023, al ricorrere delle seguenti condizioni: essere in possesso di un contratto a tempo determinato ed essere in servizio su posto vacante. Entrambe le condizioni sono soddisfatte sia nel caso di una supplenza su posto vacante disponibile (supplenza annuale, quindi, fino al 31 agosto 2025), sia nel caso di una supplenza su posto vacante accantonato appositamente ai fini dell'assunzione dei vincitori di concorso della procedura in questione; supplenza fino a nomina avente diritto e comunque con termine al 31 dicembre 2024. In ragione del preciso dettato normativo, la soluzione adottata dagli uffici scolastici regionali risulta pertanto corretta, anche alla luce della *ratio* della norma volta alla preminente salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che costituisce l'interesse primario che orienta le scelte del Ministero. Quanto all'ulteriore opzione auspicata dall'interrogante, circa la possibilità di consentire la scelta della sede per il prossimo anno scolastico già nel corso del corrente anno scolastico, si osserva che tale soluzione non risulta praticabile. Infatti, in tali casi non vi è ragione per non applicare la previsione generale contenuta all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, che prevede, per tutti i vincitori di concorso, la conferma presso la stessa istituzione scolastica ove si è svolto il periodo di prova.

luglio. Non eravate pronti e si è creato un caos che ha danneggiato sia i ragazzi e le ragazze, ma anche i candidati, coloro che erano nelle prime posizioni della graduatoria, che in servizio sono stati privati della possibilità della scelta; inoltre, gli altri vincitori non hanno potuto scegliere i posti dei confermati. Si tratta, quindi, di un quadro complessivo di caos e anche di un pasticcio che a noi continua ad apparire tale, nonostante la sua risposta. Ci sono, infatti, posti liberi su cui non si è potuto fare le assunzioni necessarie e che sono andati comunque a supplenze in attesa del nuovo concorso, mentre non si fanno scorrere le graduatorie; inoltre c'è carenza di docenti in molte Regioni per la criticità di questi posti accantonati.

quindi fortemente preoccupati e pensiamo che questo Governo stia mettendo davvero in discussione la serenità e la possibilità di avviare l'anno scolastico, come sarebbe dovuto innanzitutto ai ragazzi e alle ragazze, ma anche al personale docente.

con riguardo alle segnalate criticità della struttura penitenziaria sita in località Torre Sinello nei pressi della città di Vasto, convertita nel 2013 in casa di lavoro, il Dicastero ha provveduto ad acquisire informazioni presso l'articolazione ministeriale preposta, nonché presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il personale attualmente in servizio presso la casa di lavoro di Vasto ammonta a complessive 68 unità forza operativa, registrando una carenza di 31 unità suddivise tra i vari ruoli rispetto all'organico previsto. Le carenze maggiori si rilevano nei seguenti ruoli: ruolo degli ispettori (-4 unità), ruolo dei sovrintendenti (-6 unità) e ruolo degli agenti assistenti (-21 unità). Va innanzitutto precisato che numerose sono le iniziative assunte dal Dicastero per colmare le scoperture di organico che si registrano in tutti gli istituti di pena del Paese. Con riferimento alla carriera dei funzionari del Corpo, il 18 dicembre 2023 è stato avviato il settimo concorso per il conseguimento della qualifica di commissario, relativo al concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario, elevato a 132 posti, al cui esito si provvederà, presumibilmente entro il mese di maggio 2025, alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale in ragione delle vacanze organiche previste. Mi permetta di sottolineare che, all'esito di questo concorso, il Governo Meloni traguarderà un risultato storico: per la prima volta un istituto penitenziario sarà dotato di un comandante titolare e, per alcuni istituti più complessi, anche di un vice comandante titolare, che renderanno salda la catena di comando e permetteranno una gestione più efficace ed efficiente sia del lavoro ordinario sia delle criticità. Lo avevamo promesso e lo stiamo mantenendo: mai più comandanti a scavalco. Inoltre, in base al decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 (il cosiddetto decreto carceri), è prevista l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori. Infine, a completamento degli interventi di potenziamento del ruolo funzionari, del ruolo funzionari, è stato indetto un concorso interno per la nomina di ulteriori 60 vice commissari. Con riferimento al ruolo degli ispettori, il 5 maggio 2024 ha preso avvio il corso di formazione per la qualifica iniziale di vice ispettore relativo al concorso pubblico per 411 posti (370 uomini e 33 donne), la cui assegnazione avverrà presumibilmente nel mese di giugno 2025. All'esito, si terrà senz'altro in debita considerazione la situazione che connota il penitenziario di Vasto, destinandovi un adeguato numero di unità del ruolo. Anche in questo caso, il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto decreto carceri, ha previsto l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria per il ruolo ispettori. Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, è in corso di svolgimento un concorso interno per titoli a complessivi 583 posti (515 uomini e 68 donne). Ebbene, nell'ambito di tale procedura l'Amministrazione ha già assegnato alla casa di lavoro di Vasto cinque unità maschili. Quanto, infine, al ruolo degli agenti assistenti, segnalo che l'organico della casa di lavoro di Vasto è stato incrementato nel luglio 2023 di 10 unità complessive (otto unità maschili e due unità femminili) in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 182° e 183° corso. Questi si aggiungono a ulteriori 6 unità assegnate in precedenza nell'ambito della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni del 181° concorso. Numerosi sono gli interventi di potenziamento del ruolo agenti assistenti posti in essere da questo Governo. In particolare, il 22 luglio scorso ha preso avvio il 184° corso di formazione allievi agenti, al termine del quale, presumibilmente nel febbraio 2025, 2025, saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le esigenze della casa lavoro Vasto mediante l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo. Ad oggi è in corso di svolgimento il concorso pubblico per l'assunzione di 2.568 allievi agenti, 1.926 uomini e 642 donne; sono attualmente in svolgimento le prove di efficienza fisica e, a partire dal 2 dicembre, si svolgeranno i test psicofisici e attitudinali. Per completezza, rimarco che, in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, è stata prevista l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 agenti di Polizia penitenziaria, 500 per l'anno 2025 e 500 per l'anno 2026. Tali assunzioni straordinarie si aggiungono a quelle già autorizzate in precedenza dalla legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che ha previsto l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 unità per un totale di 2.000 extra-assunzioni finanziate da questo Governo nell'arco di un biennio. Per quanto riguarda il trattamento dei detenuti, si rappresenta quanto segue. L'istituto di Vasto ha subito nel tempo importanti trasformazioni. Recentemente, con decreto ministeriale del 23 febbraio 2023, la terza sezione internati è stata soppressa e, in luogo di essa, è stata istituita una sezione di casa di reclusione a trattamento intensificato. Tale innovazione segue una proposta di rivisitazione dei circuiti detentivi incentrata sulla tipologia di ristretti ivi presenti - internati, imputati e condannati - nonché sulle caratteristiche strutturali dell'istituto e sulle risorse di personale disponibili, elaborata dal provveditorato regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, di concerto con la direzione della casa lavoro di Vasto. Tale proposta prevedeva di destinare il terzo piano del reparto internati a sezione di reclusione, così da garantire una ripresa dei laboratori, considerato che gli internati presenti in struttura risultano affetti da patologie di tipo psichiatrico che non ne consentono un adeguato impiego in determinate attività lavorative. Quanto alle presenze di detenuti al 24 ottobre 2024 presso detta casa lavoro, erano presenti 96 ristretti, di cui cui 52 internati a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi 197 posti, di cui 50 non disponibili a causa di lavori di manutenzione ordinaria presso le sezioni prima accoglienza e reclusione a trattamento intensificato. Venendo alle attività in cui i ristretti possono essere impiegati presso l'istituto, risulta essere attiva una sartoria dove si producono federe per l'amministrazione penitenziaria, dove sono impiegati solo internati. L'istituto, peraltro, ha recentemente ottenuto 6.000 euro per il rilancio di una delle quattro serre presenti. A questo proposito, va segnalato che sono in corso sopralluoghi per valutare l'avvio di un'azienda agricola tramite cooperative esterne. La direzione sta comunque valutando anche la possibilità di una gestione diretta dell'azienda agricola, con destinazione dei prodotti delle lavorazioni a scopi solidali, in collaborazione con associazioni locali di volontariato. Sono previsti inoltre corsi a cura del CPIA di Chieti e Pescara a carattere modulare e orientamento tecnico, ad esempio scienze, arte, disegno e pittura, oltre che informatica e matematica, modulati in base alla tipologia di ristretti presenti e considerata ovviamente la presenza di internati. Infine sono attivi corsi di qualificazione professionale. La direzione dell'istituto cura poi cura poi diverse attività culturali o ricreative. Con riferimento al tema ambientale, si evidenzia che la casa di lavoro è collocata fuori dal contesto cittadino, a una distanza di circa un chilometro dal mare e a circa 600 metri dalla riserva naturale regionale denominata Punta Punta Aderci. Ebbene, a questo proposito, occorre innanzitutto precisare che tanto la predisposizione della rete fognaria pubblica quanto l'allestimento di un sistema di illuminazione adeguato sulla strada di accesso all'istituto sono evidentemente di competenza dell'amministrazione comunale. In pieno spirito di leale collaborazione istituzionale, la direzione dell'istituto si è da tempo attivata per chiedere alla predetta amministrazione comunale la realizzazione delle opere necessarie a dotare la struttura del collegamento alla rete fognaria e a migliorare la viabilità che conduce alla stessa. Ciò detto, mi preme segnalare che la struttura è regolarmente servita da un depuratore dei reflui in uscita, autorizzato con provvedimento regionale perfettamente funzionante e adeguato rispetto alla capienza dell'istituto, come accertato dalle continue ispezioni delle autorità competenti e dalla mancanza di successive contestazioni. Infatti, vengono eseguite analisi di laboratorio delle acque depurate a cadenza mensile. Inoltre, le autorità marittime preposte alla tutela dell'ambiente effettuano controlli delle acque di scarico a campione e senza preavviso. Gli esiti degli accertamenti hanno consentito di verificare il corretto funzionamento del depuratore e la conformità ai requisiti di legge. Tant'è vero che l'ultima ordinanza di interdizione temporanea alla balneabilità del tratto del mare antistante la struttura penitenziaria risale al settembre 2021. Peraltro, recentemente l'istituto ha commissionato il compimento di alcuni lavori per la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione, che prevedono un sistema di monitoraggio e telecontrollo del funzionamento in tempo reale del depuratore, attraverso l'installazione di sensori che segnalano in tempo reale eventuali anomalie.

«Report» tenutasi qualche giorno fa, che evidentemente ha aiutato a sollecitare la risposta stessa. Entrambe le interrogazioni riguardano la struttura di Vasto. Le risposte che ho ricevuto sono del tutto insufficienti. Rispetto ai numeri, se ho capito bene, ci si annuncia che da qui forse a maggio o giugno dell'anno prossimo ci sarà qualche decina di assunzioni per tutta Italia. Italia. Stiamo parlando di un istituto che ha una scopertura molto grave. Lei ha citato i 68 dipendenti che attualmente sono sono in quella casa di lavoro. Ricordo però che, di questi, 28 unità non possono essere impiegate a causa di trasferimenti o a causa di condizioni psicofisiche. Per cui da una pianta organica che è sostanzialmente di 100 dipendenti, noi abbiamo 38 A tale condizione si aggiunge un congedo ordinario accumulato dal 2019 al 2022 di circa seimila giorni. giorni. Negli ultimi giorni abbiamo letto sui giornali la fuga degli agenti penitenziari dalle nostre carceri e capiamo benissimo di che cosa stiamo parlando, e cioè di un fenomeno per il quale, rispetto ad alcune piante organiche, c'è una scopertura

ci sono state 4.500 condanne per trattamenti disumani. Tanto per fare un paragone: se nel 1990, a fronte di 3.000 omicidi, noi avevamo 25.000 detenuti, oggi, che abbiamo 300 omicidi, abbiamo 60.000 detenuti,

Questa è la condizione delle carceri nel Paese e l'abbiamo più volte denunciata. Abbiamo chiesto al Governo e chiediamo ai parlamentari di maggioranza di andarci, di svolgere questa attività, di farlo più spesso e capire direttamente che cosa succede in quegli istituti, ad esempio a Vasto: questa casa lavoro ha perso nel tempo anche la sua funzione, per cui ci sono pochissimi laboratori. Ci ha raccontato dei faremo e dei diremo, ma di fatto, allo stato attuale, abbiamo una condizione per la quale ci sono pochissime unità per decine e decine di reclusi, che sono sostanzialmente senza una prospettiva di recupero.

di una Regione che è fatta di parchi: abbiamo tre parchi nazionali, un parco regionale e decine di riserve naturali. Quella che ho citato è una delle più emblematiche, una delle più conosciute. In questo territorio, in particolare il Comune di Vasto e la sua amministrazione hanno investito negli anni moltissimo nel turismo nel turismo sostenibile, tipico di quelle zone, ossia una zona di mare all'interno di un territorio che offre moltissime esperienze di cittadinanza temporanea che riguardano tutto il suo patrimonio naturale e culturale. A fronte di questo, c'è una fossa Imhoff che viene utilizzata per lo sversamento dei liquami in mare, e oggi capisco dalla risposta che il barile viene rispedito all'amministrazione comunale. Di fatto, lì c'è il divieto di balneazione e non si può avere la sesta Bandiera blu

Capisco oggi che si chiede che questo lavoro lo faccia l'amministrazione comunale. Chiedo che davvero, nello spirito della leale collaborazione che qui viene citato, il Ministero e l'amministrazione comunale facciano un tavolo e si risolva questo problema, perché allo stato attuale è stato difficile avere una risposta anche per la stessa trasmissione che ho citato, «Report», che pure ha cercato interlocuzioni con l'istituto di pena e con il Ministero; risposta che abbiamo oggi con la frase che se ne deve occupare il Comune (non tanto nello spirito di leale collaborazione), cosa che lo stesso Comune probabilmente viene a scoprire oggi attraverso questa risposta in Parlamento. Penso che chiunque se ne debba occupare, lo debba fare presto, in leale collaborazione e risolvere il problema.

Signor Presidente, con riguardo alle criticità segnalate dall'onorevole interrogante e inerenti la carenza di organico della casa circondariale di Volterra, segnalo in apertura che la dotazione organica del reparto di Polizia penitenziaria della casa di reclusione di Volterra presenta una carenza di personale in linea con quella sofferta dagli altri istituti di pena della Nazione. Nella casa circondariale di Volterra, il personale in servizio alla data del 25 ottobre 2024 ammonta a complessive 66 unità di forza operativa, registrando, rispetto all'organico previsto, una carenza di 16 unità appartenenti ai diversi ruoli. Mi permetta di cogliere l'occasione per ringraziare gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria e del comparto funzioni centrali per l'egregio lavoro che svolgono presso l'istituto di Volterra. Lo stesso interrogante, infatti, riferisce di aver constatato l'ottimo livello delle condizioni di detenzione in tale istituto. Le carenze maggiori si rilevano nei seguenti ruoli: ruolo dei funzionari, meno due unità; ruolo degli ispettori, meno una unità; ruolo dei sovrintendenti, meno quattro unità; ruolo degli agenti assistenti, meno cinque unità. Con riferimento alla carenza di personale della carriera dei funzionari del Corpo, per integrare l'organico del predetto ruolo il 18 dicembre 2023 è stato avviato il 7° corso per il conseguimento della qualifica di commissario relativa al concorso pubblico per 120 posti di allievo commissario, elevato successivamente a 132 posti, al cui esito si provvederà, presumibilmente entro il mese di maggio 2025, alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale in ragione delle vacanze organiche previste. Mi permetta di ribadire nuovamente che, all'esito di questo concorso, il Governo Meloni traguarderà un risultato storico: per la prima volta ogni istituto penitenziario sarà dotato di un comandante titolare e, per alcuni istituti più complessi, anche di un vice comandante titolare, che renderanno salda la catena di comando e permetteranno una gestione più efficace ed efficiente sia del del lavoro ordinario, sia delle criticità. Lo avevamo promesso e lo stiamo mantenendo: mai più comandanti a scavalco. Inoltre, in base al decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carceri), è prevista l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori. Infine, a completamento degli interventi di potenziamento del ruolo funzionari, è stato indetto un concorso interno per la nomina di ulteriori 60 vice commissari. Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, segnalo che il 5 maggio 2024 ha preso avvio il corso di formazione per la qualifica iniziale di vice ispettore relativo al concorso pubblico per 411 posti (378 uomini e 33 donne). Pertanto, all'esito del citato corso di formazione, l'amministrazione penitenziaria terrà nella massima considerazione la situazione di carenza di personale che connota il penitenziario di Volterra, provvedendo all'assegnazione di un adeguato numero di unità di ruolo, che avverrà presumibilmente nel mese di giugno 2025. Si rimarca anche in questo caso che il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (decreto carceri) ha previsto per il ruolo ispettori l'assunzione di ulteriori unità mediante scorrimento della graduatoria. Con riferimento al ruolo dei sovrintendenti, evidenzio che, in esito al concorso interno per complessivi 583 posti (515 uomini e 68 donne) relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2018 e il 31 dicembre 2020 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile, l'amministrazione penitenziaria ha assegnato al reparto di Polizia penitenziaria della casa di reclusione di Volterra due unità maschili. Inoltre, è stato bandito un ulteriore concorso interno per titoli per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, per complessive 293 unità, a copertura delle vacanze delle vacanze al 31 dicembre 2022. All'esito della citata procedura concorsuale verrà tenuta in debita considerazione, anche in questo caso, la carenza del ruolo sofferta dal carcere di Volterra, con l'assegnazione di un idoneo numero di unità del ruolo. Con riferimento al ruolo agenti assistenti, segnalo che l'8 luglio 2024 hanno preso servizio negli istituti penitenziari n. 1.702 agenti (1.207 uomini e 495 donne) vincitori del concorso pubblico per 1.758, elevati elevati a 1.867 allievi agenti del 183° concorso. In tale occasione, nel mese di giugno 2024, l'organico del reparto di Polizia penitenziaria dell'istituto in esame è stato incrementato di un'unità femminile dal piano di mobilità ordinaria. Questa si aggiunge a un'altra unità maschile già assegnata a Volterra in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni del 181° corso. Numerosi sono gli interventi di potenziamento del ruolo agenti assistenti posti in essere da questo Governo. In particolare, segnalo che il 22 luglio scorso ha preso avvio il 184° corso di formazione per l'assunzione in ruolo di 1.386 agenti (958 uomini e 428 donne) che assumeranno servizio presumibilmente nel mese di febbraio 2025. Anche in questa occasione saranno debitamente

e attitudinali. Per completezza, rimarco che, in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, è stata prevista l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 agenti di Polizia penitenziaria, 500 per l'anno 2025 e 500 per l'anno 2026. Tali assunzioni straordinarie si aggiungono a quelle già autorizzate in precedenza dalla legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che ha previsto l'assunzione straordinaria di ulteriori 1.000 unità per un totale di 2.000 extra-assunzioni finanziate da questo Governo nell'arco di un biennio.

se queste assunzioni ci saranno effettivamente. Lei ha parlato di giugno 2025 e noi auspichiamo che così sarà. Nel frattempo sono state assegnate due unità di sovrintendenti, uno più uno di agenti assistenti al carcere di Volterra.

la carenza totale del personale di Polizia penitenziaria prevista si attesta al 15,85 per cento. Sono livelli piuttosto preoccupanti, anche perché quel carcere è davvero da considerare un fiore all'occhiello nel panorama nazionale:

Quando il personale è insufficiente ed è costretto a organizzarsi in qualche modo per garantire la sicurezza all'interno del carcere, tutti i trattamenti vengono perduti. Si dovrebbe quindi rinunciare alla scuola media e superiore e sarebbe

si rinunciasse a mandarvi del personale, magari distribuendolo in altre carceri dove la sicurezza è più a rischio. Se in questo carcere la sicurezza non è a rischio è perché si è investito molto anche dal punto di vista culturale e, quindi, suggerisco di non rinunciare a quanto si

Faccio sommessamente notare che, al momento, l'unico *record* che abbiamo visto in questo settore è quello delle pene e del loro inasprimento, nonché dei reati che ogni giorno vengono inventati. vengono inventati. Per tutte queste ragioni, non posso ritenermi soddisfatta, anche se auspico che si tenga in considerazione quanto oggi ho fatto osservare.

il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la sua presenza. Parliamo oggi di un tema estremamente importante che è la nostra moda, spesso nell'immaginario collettivo un luogo di lustrini, di effimero, di cose belle e voluttuarie. Invece, la moda è una colonna portante della nostra economia; per beneficio di chi ci segue da casa, parliamo di 60.000 imprese, 600.000 addetti, 100 miliardi di fatturato (forse quest'anno un po' meno, perché si sente

il vostro Governo, signor Ministro, sia legato a quell'immagine della moda come una cosa che ha a che fare col voluttuario e con l'effimero e non dia a quel settore l'attenzione necessaria. Le faccio due esempi, il primo dei quali risale ormai a qualche mese fa (io quest'interrogazione l'ho presentata nel mese di gennaio, ma non mi fu mai data risposta) e riguarda Confindustria Confindustria moda, che era la federazione di federazioni confindustriali che si erano messe insieme, facendo finalmente sistema (diciamoci la verità: uno dei problemi che abbiamo in questo nostro Paese spesso non è quello di fare le cose bene, perché le facciamo benissimo, ma di farle insieme). Ebbene, Confindustria moda aveva creato questo grande soggetto associativo dentro Confindustria, che naturalmente aveva molto più peso

questa confederazione a un certo punto si è rotta. Capisco che le associazioni imprenditoriali abbiano la loro autonomia, ma mi chiedevo cosa il Governo avesse fatto per esercitare almeno una certa *moral suasion* e tenere questo gruppo tutto insieme. Vi è un secondo esempio, forse ancora più importante, perché le nostre imprese della moda tra il 2015 e il 2019 hanno usufruito giustamente dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo per i loro campionari. Il campionario è per un'azienda di moda il prototipo, per così dire, ossia ciò che si crea per vedere vedere se poi funziona, può essere venduto e quant'altro. A un certo punto, con effetto retroattivo, si è detto: dovete restituire praticamente un miliardo di soldi già ricevuti, perché i vostri campionari non sono ricerca e sviluppo. cosa siano. Allora, se non capiamo che per un'impresa di moda il taglio, il prototipo o il nuovo tessuto sostenibile sono esattamente ciò che per un'azienda metalmeccanica è un motore o che per un'azienda tecnologica è un pezzo di innovazione tecnologica, allora vuol dire che la nostra idea della moda non appartiene al presente, ma a un passato un po' folkloristico che, secondo me, rappresenta un'ingiustizia per un settore così importante.

(in parte lo ha detto anche lui) che l'oggetto specifico della sua richiesta, riguardo alle modalità con le quali il sistema moda Italia e Confindustria moda decidono di operare, attiene esclusivamente alle relazioni tra le parti, rispetto alle quali il Governo in alcun modo può e deve interferire, anche se noi, come dimostra il tavolo della moda, lavoriamo sempre col sistema Italia nel suo complesso e cerchiamo di far lavorare tutti insieme. Colgo però l'occasione di questo *question time* per evidenziare al Parlamento quello che il Governo ha messo in atto a tutela di un settore centrale e di eccellenza del *made in Italy,* come esito anche del confronto con tutti gli operatori che abbiamo realizzato nel tavolo moda al Ministero. Un primo intervento urgente ha consentito l'estensione della durata della garanzia pubblica concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e da SACE nei casi di moratoria e ristrutturazione del debito concessa dalle banche. un'iniziativa importante, sostenuta dall'Associazione bancaria italiana, che ha diffuso anche un'apposita circolare operativa. In merito alla questione annosa del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, credo sia necessario precisare che è una pesante eredità del passato, perché deriva dalla norma poco chiara di oltre dieci anni fa e da interpretazioni che si sono susseguite in modo contraddittorio negli anni, fino alla risoluzione del 2021 (tre anni fa), che ha escluso in maniera chiara l'applicazione dell'incentivo ai campionari. Per risolvere questo grave lascito del passato, che rischia di soffocare il sistema della moda, abbiamo fatto un primo intervento per evitare conseguenze penali, prevedendo una procedura di riversamento spontaneo. Un secondo intervento lo abbiamo introdotto proprio in questa manovra di bilancio, destinando 190 milioni di euro alle imprese che hanno aderito a questa procedura di riversamento, misura che speriamo di poter migliorare a breve. Nell'ottica poi di evitare il riproporsi di complessità interpretative rispetto al nuovo credito d'imposta in ricerca e sviluppo, sono state emanate le linee guida per la corretta applicazione del beneficio. Abbiamo poi varato una misura straordinaria per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori del settore, prevedendo otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 ai lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane, con un numero di addetti pari o inferiore a quindici. Inoltre, con la legge quadro sul *made in Italy,* abbiamo messo a disposizione del settore 30 milioni per iniziative volte a sostegno dei processi di produzione di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo o comunque volti a favorire la transizione ecologica e digitale. È nostra intenzione affrontare in modo strutturale anche la questione centrale del consolidamento della filiera con interventi che favoriscano processi di aggregazione già nella prima legge annuale per le piccole e medie imprese, che presenteremo in Parlamento entro la fine di quest'anno.

formale che mi ha dato all'inizio. Sappiamo giustamente che le imprese e le loro associazioni hanno la massima libertà, ma anche che il Governo accompagna i settori produttivi, finanziandoli e sostenendoli, con missioni imprenditoriali (quando si fanno, se si fanno) e con le fiere. Il ragionamento che intercorre tra Governo e associazioni imprenditoriali consente anche di vedere situazioni di crisi quando sono proprio all'albore e al nascere e, se un Governo si interessa, non si arriva alla disintegrazione di un'associazione imprenditoriale, perché esso dovrebbe anticiparla, essere presente e sentire le parti e, quando si accorge che c'è un problema, operare subito, non dopo, dicendo che non poteva fare niente. In secondo luogo, i 190 milioni sono ben poca cosa, signor Ministro, perché, come ho detto,

autodichiarandosi colpevoli in un certo senso, alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate, tant'è che sappiamo che tantissimi imprenditori decideranno di intraprendere un'azione contenziosa nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'amministrazione finanziaria, per poter dare diritto alle loro ragioni. Si sarebbero dovuti fare un saldo e stralcio, signor Ministro, oppure una proroga, cose che le associazioni degli imprenditori hanno chiesto con grande apertura, addirittura comprando pagine di giornali. Non si può dire sempre che la colpa è di chi c'era prima e di ciò che abbiamo ereditato, perché governare significa risolvere i problemi che si presentano quando si presentano, se si è capaci di farlo. Ebbene, se non ne siete capaci, questo è fonte di grande preoccupazione per questa opposizione.

Nel 2018, l'allora ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio nominò tre

i commissari hanno ceduto il ramo *core* di Condotte assieme alla partecipazione di Eurolink a una terza società. Questa cessione è avvenuta senza una gara pubblica, probabilmente anche senza una perizia che desse una valutazione precisa della partecipazione in Eurolink,

una parcella pari a 34 milioni di euro. Capite bene che, visti i numeri della cessione di Condotte e della partecipazione del consorzio, 34 milioni di euro sembrano essere una parcella abbastanza elevata.

ma la vendita della partecipazione in Eurolink, cioè nella società che realizzerà il Ponte sullo Stretto, si è conclusa in tempi *record*, in soli quindici giorni. Nello specifico, nel breve periodo intercorrente tra l'approvazione del decreto-legge del 16 marzo e la pubblicazione dello stesso decreto-legge in *Gazzetta Ufficiale*, è avvenuta il 31 marzo. È come se il proprietario di un terreno agricolo, ormai abbandonato a pascolo, si determinasse a regalare lo stesso dopo la delibera della Giunta che lo rende edificabile a poche ore dalla sua efficacia, il giorno prima. Non basta: la vendita avviene in assenza di una gara pubblica, poiché quella svolta dai commissari non ha mai riguardato la partecipazione in Eurolink, evidentemente considerata inutile e sulla base di un valore determinato da una perizia risalente addirittura al 2021, quando il Ponte sullo Stretto di Messina era un'opera ormai del tutto accantonata. È per queste ragioni che il Ministero, dopo un'approfondita istruttoria, a novembre 2023 ha deciso di attivare la procedura per l'eventuale annullamento in autotutela dell'autorizzazione alla cessione della partecipazione in Eurolink. In quel contesto, i commissari mi hanno richiesto un incontro che, in spirito di assoluta collaborazione, ho accettato, ma che, come emerso dall'articolo citato, aveva il solo obiettivo di registrare clandestinamente le mie parole e quelle dei funzionari del Ministero. Parliamo di registrare nella stanza del Ministro. In quell'occasione, per superare le evidenti criticità già rilevate, il Ministero ha chiesto ai commissari di selezionare un consulente cui affidare l'incarico di determinare il reale valore della partecipazione in Eurolink aggiornata al momento della vendita, proponendo, sempre in spirito di collaborazione, di considerare per l'affidamento dell'incarico le maggiori società di consulenza. I commissari, invece, hanno incaricato un loro consulente, che ha valutato la partecipazione del 15 per cento in Eurolink in un *range* compreso tra un valore positivo di 4-5 milioni e addirittura un inverosimile valore negativo di 5,2 milioni. Insomma, secondo il loro consulente, la società acquirente ci avrebbe fatto un piacere a prendersi quella quota, anzi, avremmo dovuto pagarla per prendersela. A fronte di tale assurdità, il Ministero ha deciso di acquisire una propria valutazione, dalla quale è emerso che la reale valutazione della partecipazione si attesta invece in un *range* di valore ricompreso tra 14 e 43 milioni, quindi da 10 a 30 volte superiore a quanto è stata effettivamente ceduta. Peraltro, un valore simile si ritrova anche nella procedura di concordato preventivo della società CMC di Ravenna, che ha realizzato, come doveroso, un'asta pubblica, con una base di almeno 11,3 milioni di euro per una quota del 13 per cento, cioè inferiore a quella di Condotte. C'è di più: a fronte di una condotta professionale a dir poco discutibile, i commissari hanno presentato una richiesta di compenso di oltre 11 milioni di euro a testa, comprensivo di quanto già ricevuto a titolo di acconto: una cifra oltre tre volte superiore al compenso spettante, in base ai parametri fissati dal decreto ministeriale del 2016, come risulta dalle istanze inviate dai commissari al Ministero il 4 luglio scorso. Se la matematica non è opinione, parliamo di una richiesta complessiva di 34 milioni di euro per un bene svenduto senza gara. Avevo quindi il dovere di intervenire a tutela dell'interesse dello Stato.

molto gravi e devono portare a valutazioni serie e puntuali, perché quanto è successo grida veramente vendetta e deve avere una valutazione seria e precisa. Innanzitutto, registrare all'interno di un ufficio del Ministro è di per sé un reato molto pericoloso e grave.

che avrebbe dato il giusto valore. Se 11,5 milioni è il valore di una partecipazione inferiore a quella di Condotte, vuol dire che la valutazione di quella in Eurolink era ben superiore a quella a cui è stata valutata e venduta

*(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, torno anch'io sulla questione di Condotte. Abbiamo appreso da un articolo del quotidiano «Domani» del 26 ottobre che sono state realizzate registrazioni clandestine nel corso di due riunioni presso il suo Ministero; erano riunioni con i commissari straordinari di Condotte d'Acqua SpA, una società in amministrazione straordinaria su cui ha specifiche competenze il suo Ministero. Nella stanza di un Ministro della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni, qualcuno avrebbe illecitamente registrato il contenuto delle riunioni per poi fornire tali registrazioni a un quotidiano, con lo specifico intento di arrecare danni all'azione del Ministro stesso: anche perché il ministro Urso sta riportando ordine e legalità nel settore delle amministrazioni straordinarie. peraltro notizia di queste settimane che nel nostro Paese operano gruppi organizzati per la realizzazione di attività illecite di dossieraggio a danno dei vertici dello Stato e di personalità politiche e della società civile. Abbiamo anche appreso, signor Ministro, da sue recenti dichiarazioni, che quando lei ricopriva il dedicato incarico di Presidente del Copasir avrebbe subito accessi illeciti alla sua corrispondenza e sui conti correnti bancari, fatti che ha puntualmente denunciato alla magistratura. Come risulterebbe dagli atti della procura della Repubblica di Perugia, nelle cui indagini risulta coinvolto Giovanni Tizian, uno dei firmatari dell'articolo del costui e altri suoi colleghi del medesimo quotidiano avrebbero ricevuto illecitamente documentazione dall'indagato Striano. Uno dei commissari straordinari, il professor Giovanni Bruno, è già salito agli onori della cronaca per vicende poco limpide, legate alla sua nomina come commissario straordinario di Eldo (società anch'essa in amministrazione straordinaria), oggetto di indagine da parte della procura di Roma, e agli strani sorteggi correlati alla sua nomina come commissario di Condotte d'Acqua, nonché agli intrecci con professionisti cui sono stati attribuiti gli incarichi di consulenza. Le chiedo quindi, signor Ministro, se le circostanze riportate risultino rispondere al vero e come intenda proseguire nell'opera di rigore e di coordinamento nella gestione della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in modo specifico, di quella di Condotte d'Acqua, nonostante gli ostacoli che le vengono frapposti.

tenutesi presso il Ministero, da me presiedute nella mia stanza, sono state oggetto di registrazione clandestina. Quello che è accaduto è di una gravità inaudita, che viola le fondamenta dell'esercizio del principio democratico affidato ai corpi dello Stato, che non devono temere di essere spiati mentre esercitano il loro mandato. L'episodio peraltro si inserisce in un contesto inquietante, come emerge da recenti inchieste giudiziarie a Perugia, Milano e Roma, che devono far riflettere quest'Assemblea. Io stesso peraltro ho dovuto constatare che, anche nel mio precedente e delicato incarico istituzionale quale Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ero stato oggetto di attenzione. Nell'agosto del 2022 ho già subito un'intrusione con l'esfiltrazione di *mail* dalla mia posta elettronica, ai fini di predisporre una gravissima azione di dossieraggio, peraltro alla vigilia della campagna elettorale (atto che denunciai subito alla procura della Repubblica). Ho inoltre appurato nell'indagine di Perugia che, nello stesso periodo ed anche in precedenza, il dottor Striano ha fatto accesso al mio conto corrente bancario. C'è da chiedersi per conto di chi l'abbia fatto per conto di chi abbia controllato chi aveva il compito, su incarico di questo Parlamento, di controllare. Cari colleghi, episodi di questo tipo minano la sicurezza dei rappresentanti dello Stato e indeboliscono l'efficacia dell'azione pubblica. Abbiamo il dovere di intervenire, come sta facendo il Governo, per rafforzare la protezione delle informazioni e prevenire interferenze indebite nella vita istituzionale. In merito a Condotte SpA, si tratta di due registrazioni clandestine, le cui trascrizioni sono state peraltro depositate dagli stessi commissari nel giudizio amministrativo in queste ore all'esame del Consiglio di Stato. Esse Esse comunque confermano in modo inoppugnabile la correttezza e la trasparenza dell'operato del Ministero, cui i commissari non hanno evidentemente corrisposto eguali trasparenza e buona fede perché non solo hanno venduto senza gara la quota di partecipazione di Eurolink, ma hanno addirittura registrato in modo fraudolento nella stanza del Ministro. Peraltro, dagli articoli citati dall'interrogante era già emerso proprio nel passato, in più occasioni, un intreccio un intreccio davvero inquietante in merito alla vicenda di Condotte, sul quale credo sia necessario fare chiarezza, anche alla luce dell'ultimo gravissimo episodio. Questo però non ci farà deflettere dall'azione di moralizzazione che abbiamo già intrapreso in merito alle amministrazioni straordinarie. Proprio nella manovra di bilancio è previsto un collegato che si ripropone di rendere più efficace l'esercizio dei poteri di vigilanza e successivamente - come ho già annunciato in Commissione alla Camera un mese fa - realizzeremo una riforma organica dello statuto delle amministrazioni straordinarie. Noi non ci facciamo intimidire, noi non siamo condizionabili. Ministro Urso, sono soddisfatto e rasserenato dalla sua risposta. Vada avanti nell'opera di garantire la miglior amministrazione per le aziende in crisi. Noi non ci facciamo intimidire. D'altro canto - lo sappiamo bene noi di centrodestra - da quando Berlusconi ha fondato l'alleanza di centrodestra, trent'anni fa, c'è sempre stato qualcuno che ha cercato di fermare la nostra azione politica con mezzi e mezzucci. Il nostro modo di governare però, con onestà e competenza, ha superato sempre gli ostacoli, non sempre leciti, che ci hanno messo davanti. Gli italiani lo sanno e continuano a riconoscercelo anche nelle urne. Buon lavoro, Ministro.

Signor Ministro, non dovrebbe esserci bisogno di riassumere con lei la situazione di crisi in cui si trova il settore dell'*automotive* in Europa e in Italia: una contrazione della produzione senza precedenti; Volkswagen annuncia la chiusura di tre stabilimenti; Stellantis rischia di finire l'anno con meno di 300.000 auto prodotte e non dà certezza sul piano dei progetti industriali; la Cina è sempre più protagonista sul mercato globale grazie al vantaggio competitivo sull'elettrico, controllando il 75 per cento della produzione mondiale di batterie. con lo stop al progetto di Termoli, continuiamo a non avere nemmeno una *gigafactory*, mentre i costruttori europei si muovono dentro orizzonti temporali ristretti e in modo non coordinato.

può pensare di fare quello che ha deciso di fare il Governo e che lei ha avallato o subìto (e, in quel caso, una riflessione da parte sua sarebbe più che mai opportuna). Ad ogni modo, non si pretendeva nemmeno uno sforzo progettuale da parte vostra. Bastava non fare danni, mantenere quello che già c'era e non toccare il fondo *automotive* istituito dal Governo Draghi per il sostegno e la promozione della transizione verde, della ricerca

(Confindustria, le principali associazioni di categoria, i tre sindacati confederali che infatti hanno organizzato uno sciopero sacrosanto il 25 ottobre scorso), con la manovra di

chiediamo di fermarvi, di rendervi conto di quanto sia scellerata questa decisione, di ripristinare le risorse e invertire la marcia il più presto possibile. Non solo: diteci che iniziative volete intraprendere a livello europeo per favorire la creazione di grandi *player* industriali. Ancora, vi attiverete per prorogare la cassa integrazione straordinaria per il settore *automotive*? Rafforzerete le politiche di sostegno necessarie alla transizione e all'evoluzione tecnologica rispetto all'elettrico? Garantirete misure di vantaggio per sostenere, nell'immediato, la domanda di autoveicoli? In assenza di tutto questo, continuerà ad avere ragione chi, come noi, pensa che questo sia un Governo a zero politiche industriali e zero crescita. Soprattutto, in assenza di risposte, le conseguenze più gravi ricadranno su un settore che rappresenta oltre il 5 per cento del PIL nazionale, sulla nostra economia e su centinaia di migliaia di lavoratori

l'Italia, né solo Stellantis, ma coinvolge l'intera industria europea, come dimostrano i drammatici annunci di chiusura di stabilimenti che si susseguono uno dopo l'altro, con conseguenti licenziamenti in blocco in tutta Europa. È urgente un intervento in Europa che riveda le regole del *green deal*, come abbiamo detto sin dall'inizio della legislatura anche in quest'Aula e come oggi chiede lo stesso Mario Draghi nel suo *report* sulla competitività. Per questo, abbiamo concordato con la Repubblica Ceca un *non paper* che chiede di anticipare a inizio 2025 la clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, che ho personalmente illustrato in queste ore agli altri colleghi europei per avere anche il loro consenso. Il documento non mette in discussione l'obiettivo della decarbonizzazione al 2035, ma chiede di raggiungerlo con un approccio di neutralità tecnologica e non gravando da subito con multe che in questa fase di transizione sarebbero un'ulteriore zavorra competitiva per i produttori europei. È una follia quella che vi descrivo. Per rispettare i *target* emissivi imposti dall'attuale regolamento ed evitare un salasso stimabile in 17 miliardi di euro già nel prossimo anno, i produttori di auto europei stanno riducendo i volumi produttivi, chiudendo le fabbriche e licenziando gli operai e, come fa Stellantis, importano e commercializzano auto elettriche prodotte in Cina per venderle nella propria rete e superare quei parametri. Due follie! Gli uni chiudono le fabbriche per ridurre la produzione, scendere sotto i parametri e non pagare le multe, gli altri importano auto elettriche, le certificano e le vendono alla propria rete di vendita per evitare di pagare le multe. La decarbonizzazione non deve portare alla desertificazione industriale; dobbiamo cambiare subito, non c'è più tempo da perdere, siamo al collasso dell'industria dell'auto europea. Sul fronte nazionale registro che le mozioni approvate da tutte le forze parlamentari alla Camera hanno dato evidenza di coesione e unitarietà di intenti, nonché di piena consapevolezza dell'urgenza del tema. La prossima settimana, il 14 novembre, si riunirà il tavolo Stellantis e ci attendiamo risposte concrete da parte dell'impresa sul destino degli stabilimenti italiani e dei lavoratori. Nel frattempo, siamo impegnati a definire nuovi strumenti di sostegno alla componentistica, la vera forza del *made in Italy*, che auspichiamo di poter annunciare già in quell'occasione. Interverremo anche in legge di bilancio per incrementare le risorse destinate alla filiera e ai processi di riconversione produttiva. Gli incentivi destinati all'acquisto non hanno avuto effetti positivi sulla produzione. Dobbiamo prenderne atto e concentrare le risorse sugli investimenti. È finito il tempo dei *bonus*. Proprio ieri ho firmato un provvedimento che prevede l'apertura del nuovo sportello dei contratti di sviluppo, finanziato con risorse del PNRR, dedicato alle filiere strategiche nazionali, includendo tra queste il settore auto. La dotazione finanziaria di 500 milioni potrà essere integrata per far fronte alle esigenze del settore nel prossimo biennio 2025-2026. Dal 2027, infatti, come previsto in legge di bilancio, è stato istituito un fondo strategico che consentirà di alimentare gli strumenti agevolativi con una dotazione complessiva di 24 miliardi nel periodo 2027-2036. La legge di bilancio, inoltre, ha creato il presupposto per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la proroga, per l'anno prossimo, della cassa integrazione straordinaria nell'ambito del settore *automotive*. Insieme, anche in Europa, dobbiamo cambiare il *green deal* per rendere sostenibile l'industria dell'auto e, in generale, l'industria europea.

non ci venga di nuovo a raccontare la storiella del *green deal*, perché oggi è in crisi l'auto, poi domani la crisi sarà ancora più grave. Sa perché oggi è in crisi, ministro Urso? Ci sono 500 auto ogni mille abitanti: lo abbiamo mai fatto questo dibattito in Aula?

la reinterpretazione della mobilità urbana, TPL, *car pooling*, ciclabili; li avete rapporti con i ragazzi di oggi? Non chiedono di acquistare l'auto, anche perché costa tanto. Abbiamo discusso o no delle ragioni dell'incremento dei prezzi, signor ministro Urso, in quest'Aula, in una mozione magari unitaria che non c'è stata, perché non vi siete mai messi nella condizione di accettare le proposte dell'opposizione?

agli incentivi all'acquisto, come lei sa, ma andavano alla ricerca, agli investimenti, alla transizione verde; anche agli incentivi, oltre che alle rottamazioni. Di quei 4,6 miliardi, i 700 milioni a cui fa riferimento Giorgetti che lei richiamava in maniera indiretta qui sono una cosa. La richiesta che ha fatto il Partito Democratico, cioè di andare non solo sulla domanda ma sull'offerta, imponeva una discussione sulla politica industriale, che lei non ha mai fatto. Signor Ministro, noi ribadiamo un tema semplice, che è nella nostra interrogazione e che il senatore Martella ha richiamato poco fa: chiediamo una discussione in sede europea sull'integrazione, sull'aggregazione, sulla capacità di avere una catena del valore comune, che consenta ai grandi marchi europei di avere una visione comune. Se manca questo la nostra accusa di un Governo che va avanti a fari spenti e che non ha la politica industriale come prima missione diventa fin troppo evidente, anche dal confronto di oggi in questo *question time.*

Signora Presidente, signor Ministro, l'interrogazione fa riferimento alla situazione di inquinamento del torrente Solofrana, storicamente affetto da problemi ambientali legati al rilascio di reflui dalle industrie conciarie. Nonostante l'esistenza di impianti di depurazione nel territorio, la contaminazione, in particolare quella da tetracloroetilene, continua a persistere, per la protezione ambientale (ARPA) Campania. Più precisamente, per quanto riguarda la matrice suolo e relativamente ai campioni di acqua sotterranea, il sito della falda profonda Solofrana-Montorese risulta potenzialmente contaminato di contaminazione (CSC) per il tetracloroetilene. Diversi studi hanno associato l'esposizione cronica al tetracloroetilene ad un aumento del rischio del cancro e pertanto il composto è stato classificato come possibile cancerogeno dall'Agenzia Il depuratore di Solofra è gestito da Cogei srl e la giunta comunale di Solofra prevede la riorganizzazione del servizio idrico e il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione a una nuova società mista Consorzio con maggioranza comunale e minoranza di imprenditori privati del settore conciario. Si evidenziano preoccupazioni riguardo ai potenziali conflitti di interesse, in quanto le aziende conciarie sarebbero coinvolte nella gestione del depuratore che tratta i loro stessi reflui, e alla necessità di non far pagare agli incolpevoli cittadini contribuenti un'eventuale bonifica. Si richiedono pertanto chiarimenti sui seguenti tre aspetti: se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali imminenti misure di competenza intenda adottare per vigilare e risolvere le succitate criticità; se ritenga opportuno applicare il principio europeo e nazionale di chi inquina paga, mediante la ricostruzione delle responsabilità in merito ai fenomeni della possibile contaminazione della falda profonda Solofrana-Montorese e se, alla luce dell'eventuale necessità della bonifica e delle ingenti risorse a tal fine indispensabili, il Ministro non ritenga necessario rivalutare la perimetrazione del sito da regionale a nazionale.

come ricordato dall'interrogante, attualmente né il Comune di Solofra, né l'area del torrente Solofrana sono ricompresi in area sito di interesse nazionale (SIN), né risultano essere indicati tra i siti orfani. Per un'eventuale individuazione futura dell'area quale SIN si rammenta che, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. la perimetrazione di un SIN viene effettuata d'intesa con la Regione interessata, secondo regole precipue e al ricorrere di condizioni prestabilite, anche relative alla perduranza sui luoghi interessati dello svolgimento di specifiche attività produttive. produttive. In merito all'accertamento del danno ambientale, le strutture competenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possono certamente attivarsi, ma solo previa segnalazione, ad oggi mai pervenuta. Data la rilevanza del tema, il MASE si è attivato per richiedere agli enti territoriali interessati di fornire elementi in merito alla sussistenza di eventuali profili di danno o minaccia di danno ambientale. Si evidenzia, ad ogni modo, che l'accertamento dell'eventuale responsabilità per la possibile contaminazione della falda profonda, in applicazione del principio europeo e nazionale del chi inquina paga, è in capo alla Provincia competente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 244 del testo unico ambientale, in questo caso la Provincia di Avellino. Nell'ottica di mantenere comunque un quadro conoscitivo in ordine alle diverse realtà di cui si compone il servizio idrico in Italia, si rammenta, come peraltro già indicato dall'onorevole interrogante nell'interrogazione, che al Comune di Solofra, in deroga alla disciplina ordinaria, con delibera del comitato esecutivo dell'ente idrico campano del 29 giugno del 2022, è stata concessa la gestione del servizio in forma autonoma, essendo stati riconosciuti i presupposti per la cosiddetta salvaguardia rispetto all'organizzazione in ambiti territoriali ottimali.

perché rileva una preoccupante sottovalutazione della gravità della situazione ambientale che colpisce quest'area. Non possiamo permetterci di considerare questa problematica come una mera questione regionale. Stiamo parlando di una delle aree più industrializzate del Paese, fortemente caratterizzata da attività conciarie che, come dimostrano i 12 sequestri di aziende avvenuti negli ultimi tre anni, hanno generato un inquinamento che non si può ignorare. I cittadini vivono quotidianamente incertezze riguardo ai rischi per la salute legati all'inquinamento ambientale e il *dossier* «Buone e cattive acque» di Legambiente segnala che, su 16 punti monitorati del bacino idrografico del fiume Sarno, ben 10 hanno una qualità insufficiente. Pertanto, è inaccettabile che il Governo - lei, Ministro - non abbia ancora designato quest'area come sito di interesse nazionale. Non possiamo permetterci questa assurdità, signor Ministro, come ha sottolineato anche la Corte dei conti europea, che ha ribadito il principio chi inquina paga, e questi non devono essere i cittadini. Ministro, la invito ad una misura coraggiosa da parte sua, ossia a dichiarare quest'area sito di interesse nazionale.

danni ingenti e anche una vittima. Le aree colpite sono quelle di Bologna, Modena e Reggio-Emilia e purtroppo i danni sono stati rilevanti: 3.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, 15.000 abitazioni senza elettricità. Provengo da una parte del territorio toscano che dal 23 settembre al 25 ottobre scorsi, è stato colpito da ben tre circoscritti fenomeni atmosferici di eccezionale rilevanza

sono state portate avanti dalle Regioni relativamente alla prevenzione del rischio idrogeologico e la gestione delle acque, in ragione di ben precise competenze che le Regioni hanno, con strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione del rischio ambientale. La domanda che le rivolgiamo, signor Ministro, è appunto quali siano gli atti che codesto Ministero intende mettere in atto per contrastare il rischio idrogeologico, incluso l'accertamento dell'effettiva attuazione da parte delle autorità regionali e locali interessate delle misure di prevenzione utili a prevenire e a monitorare tali eventi e a salvaguardare anche la vita delle persone.

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che per la definizione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (stralcio 2024), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha messo a disposizione di Regioni e Province autonome risorse di bilancio per circa 1.084 milioni. Sono attualmente in corso le attività amministrative finalizzate alla definizione del suddetto Piano, di cui si prevede la conclusione entro fine anno. Come è noto, il dissesto idrogeologico è uno dei temi affrontati dal decreto-legge ambiente - ora all'esame di questo ramo del Parlamento - che reca una pluralità di disposizioni volte a rendere più efficace e tempestivo il sistema integrato di monitoraggio degli interventi di difesa del suolo e più snella la programmazione delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, oltre al monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, a partire dalla piattaforma ReNDiS, che mira a garantire che tutti i livelli di governo possano disporre di un quadro conoscitivo indispensabile per presidiare la realizzazione di interventi di così elevata rilevanza, anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari. L'attuazione degli interventi di cui si compone il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico resta affidata ai presidenti delle Regioni, in veste di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, i quali, tra l'altro, sono responsabili del corretto e tempestivo inserimento dei dati nei sistemi di monitoraggio dedicati e sono altresì tenuti a relazionare con cadenza annuale sullo stato di attuazione degli interventi. Sulla base di tali dati, il Ministero redige la relazione contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. La relazione del 2024, contenente i dati aggiornati al 31 dicembre scorso, è in fase quindi di completamento. Si conferma l'attenzione di questo Dicastero, per quanto di competenza naturalmente, sul tema in oggetto, senz'altro meritevole di essere gestito all'unisono con gli uffici del Ministero e della Protezione civile sulla base di un quadro chiaro utile tanto nella fase di prevenzione quanto in quella emergenziale, ricordando peraltro che su questi temi intervengono anche altri Ministeri, quali il Ministero dell'interno, in un suo ribaltamento sui Comuni, e il Ministero delle infrastrutture per quanto riguarda le opere; è quindi sempre necessario un concerto.

il dubbio che in due Regioni, Emilia-Romagna e Toscana, i rispettivi Presidenti non abbiano fatto bene il loro lavoro o non lo abbiano certamente tenuto in debita considerazione, come questo Governo invece ha fatto attraverso misure importanti, quali il decreto-legge n. 61 del 2023, rivolto a una serie di misure per mitigare gli effetti di questi cataclismi atmosferici e, ancora e ancor di più, il decreto-legge n. 76 del 2024, con il quale siamo andati addirittura a introdurre delle agevolazioni utili per l'acquisto di aree alternative per l'edificazione, evidentemente in sostituzione degli edifici Quindi mi sento di poter rassicurare anche i miei concittadini sui territori di Livorno e di Pisa, pesantemente colpiti nelle scorse ore da questi fenomeni, e la ringrazio a nome del Gruppo Lega.

il mercato del lavoro appare ormai in una fase di consolidato rilancio, come testimoniato dai dati Istat, che anche nell'ultima rilevazione, pubblicata il 31 ottobre 2024, attestano un numero di occupati ormai stabilmente intorno alla soglia dei 24 milioni di unità. In questo contesto residuano ancora alcuni comparti produttivi in cui si avvertono significative difficoltà nel reperimento di personale, dovute a diversi fattori, tra cui la tendenza demografica negativa. Oltre a proseguire nel rilancio della formazione professionale e nel processo di riduzione del *mismatch* interno alla domanda e offerta di lavoro, appaiono utili politiche migratorie in grado di garantire l'ingresso nel Paese di ulteriori lavoratori opportunamente formati. Le politiche adottate nell'ultimo biennio, in controtendenza con il recente passato, si sono opportunamente caratterizzate per aver privilegiato flussi migratori regolari, pianificati a monte attraverso una programmazione strutturata. Con il decreto-legge flussi 2023-2025, infatti, si è per la prima volta elaborata una programmazione dei flussi su base triennale (2023-2025). Il decreto-legge n. 20 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2023, ha inoltre posto al di fuori delle quote di ingresso i cittadini stranieri che completano programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La promozione dell'immigrazione regolare risulta altresì funzionale a garantire che i lavoratori siano effettivamente tutelati e protetti, ponendosi come ulteriore strumento indiretto di contrasto al caporalato e al lavoro sommerso irregolare. Coerentemente con questa visione, il decreto-legge n. 145 del 2024, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevede, accanto a disposizioni di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori di ingresso in Italia per motivi di lavoro. In questo scenario appare fondamentale la collaborazione con i Paesi dell'area mediterranea, promuovendo progetti che garantiscano prepartenza ai lavoratori e un'adeguata formazione tanto sul fronte professionale quanto su quello linguistico e sugli aspetti di sicurezza del lavoro. Si chiede di sapere quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per implementare la collaborazione con i Paesi dell'area del Mediterraneo, soprattutto al fine di favorire progetti volti alla formazione qualificata dei lavoratori nell'ambito della più ampia strategia di promozione dell'ingresso regolare di stranieri in Italia.

nello spirito della Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo che si è svolta a Roma a luglio 2023 e del vertice Italia-Africa del 29 gennaio di quest'anno. Da questi impegni importantissimi è scaturito il Piano Mattei, che risponde all'interesse di creare un nuovo modello di sviluppo e partenariato con l'Africa. Uno dei pilastri su cui il Piano Mattei si fonda è la promozione di attività di formazione in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, anche attraverso l'attivo coinvolgimento delle imprese. L'obiettivo dell'effettivo e tempestivo impiego dei lavoratori stranieri è perseguito dal nuovo decreto flussi, il decreto-legge n. 145 del 2024, laddove si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Allo stesso scopo sono dirette altre norme previste nel decreto flussi quali, a titolo esemplificativo, la disposizione che stabilisce che, entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno. La norma, inoltre, pone particolare attenzione proprio sulla formazione all'estero. È confermata la previsione che la frequenza di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi d'origine consente ai lavoratori stranieri formati di arrivare in Italia al di fuori delle quote dei decreti flussi. I corsi possono essere promossi da vari attori, come le Regioni e le parti sociali, gli operatori del mercato del lavoro e gli enti di formazione, anche in partenariato. Attualmente il Ministero ha approvato venti progetti, di cui sette coinvolgono i Paesi dell'area del Mediterraneo, con una particolare attenzione verso i Paesi del Sud del Mediterraneo. Tra questi, la Tunisia è indubbiamente in questo momento il *partner* principale. A questo proposito, il Memorandum d'intesa del 20 ottobre 2023, siglato con il Governo tunisino, rappresenta un passo significativo per il rafforzamento dei canali legali di immigrazione. Nel caso specifico della Tunisia, sono stati approvati finora tre progetti, che riguardano il settore dell'edilizia, oltre che il settore navale e quello agricolo. Nel corso della missione del 4 novembre scorso a Tunisi, ho rinnovato alle autorità di governo locali il nostro impegno a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale, avviando un corso di formazione in materia edile denominato Thamm Plus, nonché l'iniziativa Global Skills Partnerships, supportata dalla Banca mondiale, destinata a dare nuovo impulso alle iniziative di formazione in corso tra i nostri Paesi. Il programma Thamm Plus, finanziato dalla Commissione europea e cofinanziato dal nostro Ministero dell'interno, in particolare ha come obiettivo la formazione, ai fini del successivo inserimento nel mercato del lavoro italiano, di 2.000 addetti al settore dell'edilizia, da formare in Tunisia, e di 500 addetti al settore della meccatronica, da formare in Marocco. Ho inoltre promosso, unitamente al mio omologo tunisino, il primo Forum italo-tunisino sulle competenze professionali e il lavoro, che è stato anche l'occasione per l'avvio di progetti sostenuti dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sulla formazione professionale in Tunisia. Continuiamo e continueremo a operare per sostenere le richieste del mercato del lavoro, garantendo, allo stesso tempo,

nel solco tracciato dal Governo per quanto riguarda i rapporti con il continente africano nei prossimi anni. È un indirizzo molto forte quello che ha dato il Governo,

ma con tutto il continente africano, in modo tale da qualificare e rendere ancor più appetibile il nostro territorio, in forma assolutamente legale, facendo arrivare persone che hanno

sul continente africano, anzi di massima collaborazione; il fatto di poter puntare sulla formazione del personale penso che sia uno degli aspetti più importanti e fondamentali per quanto riguarda il piano.